parere non ostativo sugli emendamenti 4.0.600 (testo 2), 4.0.601, 4.0.602 e 4.0.610. La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.0.1 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

prevedendo l'utilizzo di 5 milioni sul fondo della meccanizzazione e 5 milioni sul fondo di solidarietà in agricoltura. Con queste modifiche, il relatore esprime parere

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione agricola, al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito derivante dalla malattia fungina Peronospora della vite (Plasmopara viticola), si provvede per l'anno 2008 per 20 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, e successive modificazioni, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato

Accetto la riformulazione del relatore nella consapevolezza comunque che questa cifra non risolve interamente il problema da me esposto, anche se costituisce significativo intervento di questo Governo sull'argomento. Sono certo che anche il Ministro dell'agricoltura che, alcuni giorni fa, commentando l'esito della campagna vitivinicola 2008, si dichiarava soddisfatto per gli incrementi di produzione riscontrati soprattutto in Sicilia, che lui quantificava nel 35 per cento, fosse assolutamente consapevole del fatto che questo incremento

al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito derivante dalla malattia fungina Peronospora della vite (Plasmopara viticola), si provvede per l'anno 2008 per 20 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, e successive modificazioni, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato e 5 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 luglio 2004, n. 102.

al solo fine di rendere il lavoro della Presidenza utile, il testo sul quale sono autorizzato esprimere il parere, *ex* articolo 100 del Regolamento, perché questo è il testo che abbiamo esaminato, è il seguente (lo leggo per intero solo perché sia chiaro quello su cui la Commissione bilancio ha discusso): «Con riferimento al Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione agricola, al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito derivante dalla malattia fungina Peronospora della vite (Plasmopara viticola), si provvede per l'anno 2008 per 10 milioni di euro, dei quali 5 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 1966, n. 910, e successive modificazioni, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato e 5 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 luglio 2004, n. 102».

che vengono reinseriti soltanto 10 milioni di euro, che non bastano a dare le risposte che servono per questo tipo di patologia che ha purtroppo colpito la viticoltura italiana. Midomando come si potrà

Ha usato un termine un po' troppo impegnativo quando ha parlato di «significativa soddisfazione». C'è poco di significativo in questo emendamento. Volevo ricordare

cresciuto senza il classico assistenzialismo che in Sicilia ha prodotto soltanto danni. È un settore innovativo

che in Sicilia, e in particolare nella Provincia di Trapani, ha espresso delle punte di eccellenza riconosciute sul mercato mondiale con premi, capacità produttive ed inedite capacità di commercializzazione del prodotto. Il Governo Prodi e la maggioranza di centrosinistra, con un contributo ampio in quest'Aula, diedero una risposta seria, senza tutti questi balletti e passaggi mortificanti che ci richiamano ad un vecchio modo di fare legislazione e politica nei confronti della Sicilia e del Mezzogiorno. L'impressione onesta di molti senatori sarà quella di ritenersi di fronte al solito intervento assistenziale, alla solita manfrina,

sono moderni, sono capaci di misurarsi con le sfide del mercato. Risolvere questa vicenda con una semplice mancia, con una semplice mancia, cercando i titoli dei giornali, non è serio né rigoroso. Ecco perché c'è poco da essere soddisfatti. Ecco perché denunciamo

Il Mezzogiorno che vuole cambiare viene mortificato. Al Mezzogiorno vecchio, invece, quello ancora ancorato alle vecchie pratiche assistenziali e clientelari, si fa l'occhiolino. Vogliamo prendere le distanze da questo modo di fare e vogliamo dire chiaramente al settore vitivinicolo che noi avanziamo proposte serie. Lo abbiamo dimostrato quando eravamo al Governo e lo continueremo a dimostrare dall'opposizione, sottraendoci a questo modo sbagliato di rispondere alle loro legittime esigenze.

la questione sollevata dal senatore D'Alì è estremamente grave per la Sicilia. Non si tratta di un provvedimento assistenziale. Probabilmente, i colleghi che non vivono la realtà climatica, microclimatica, ambientale della Sicilia non comprendono cosa significhino venti sciroccali, peronospora, sabbia vulcanica, cosa significhino

in futuro. Un ragionamento di questo genere non può essere fatto in questo momento, ma non è da escludere - anzi è da auspicare - che la Commissione agricoltura dedichi

Grazie,

Signora Presidente, cari colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, il decreto-legge in esame si propone di completare un percorso legislativo già avviato ai fini di intervenire a sostegno dell'agricoltura, un ramo della nostra economia importantissimo che sta attraversando un periodo molto difficile e questo settore, in Regioni di montagna come la mia, la Valle d'Aosta, è ancora più in difficoltà. Sin dalla sua originaria impostazione, il decreto prevede disposizioni in materia di promozione del settore agroalimentare italiano all'estero, intervenendo sullo strumento del credito d'imposta della legge finanziaria 2007. La modifica a questa norma della finanziaria 2007 si rende urgente in quanto, dopo un complesso negoziato, la Commissione europea, con decisione del 13 febbraio 2008, ha approvato lo schema di decreto attuativo del regime di aiuti in questione. Esso si propone inoltre di disciplinare l'assegnazione del contingente di biodiesel defiscalizzato per i restanti anni di validità del programma pluriennale di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, Anche tale misura si è resa necessaria per consentire alle imprese operanti nella filiera del biodiesel di poter programmare i contingenti di biodiesel in anticipo rispetto alla scadenza dell'agevolazione fiscale. Si prefigge ulteriormente di risolvere un'emergenza di carattere finanziario e gestionale correlata ai tempi e alle procedure contabili nazionali ed europee, inerenti agli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'agricoltura. Spero che questi traguardi possano essere raggiunti, ma non ritengo che il provvedimento in esame risponda a quei carattere di sistematicità e organicità che la materia richiede. In tal senso, mi preme sottolineare l'importanza, come previsto dalla cosiddetta legge Alemanno, dell'applicazione degli sgravi di natura contributiva fiscale a favore delle zone svantaggiate e montane comprese nell'Obiettivo 1. Altrettanto urgente ritengo - in un momento in cui la questione energetica è al centro dell'attenzione non solo nazionale ma mondiale, in materia di bioenergia l'applicazione delle relative norme di attuazione. La grave crisi che il settore agroalimentare sta attraversando necessita di interventi di tipo strutturale, che non andrebbero adottati con provvedimenti emergenziali. Ci auguriamo, quindi, che si possa pervenire ad una adeguata sistematizzazione del settore agroalimentare nel disegno di legge governativo, presentato dal Consiglio dei ministri il 31 ottobre 2008. Nel frattempo facciamo appello anche al Governo affinché non solo si esprima ma riveda i tagli previsti in finanziaria. Al riguardo l'aver approvato l'emendamento 1.0.1, limitato nel tempo per mancanza di fondi, sottolinea la correttezza della richiesta ma dall'altra parte la mancanza di fondi per questo settore. In questa fase di acuta crisi economica il settore agricolo non può permettersi tagli indifferenziati ed un'ulteriore riduzione di risorse, come non può accettare provvedimenti dettati per tamponare esigenze immediate, ma richiede una revisione complessiva. Il Governo dovrebbe piuttosto abbattere gli oneri burocratici che soffocano questo settore. Auspico che l'Esecutivo si mostri sensibile alle questioni da noi sollevate, dimostrando di tenere davvero ad un settore portante della nostra economia, che non può essere abbandonato, specie in un periodo nel quale una vasta crisi economica su scala mondiale sta colpendo tutti, dalle famiglie alle piccole e medie imprese.

voglio solo spiegare i motivi del nostro voto contrario a questo decreto, visto che siamo partiti in Commissione con un clima, come ho detto ieri, costruttivo:

Lo abbiamo fatto con molta attenzione e decisione, perché ci crediamo, perché l'Italia dei Valori crede - ripeto - che solo con l'agricoltura e sopratutto nel Sud possiamo dare quella ripresa e quello sviluppo economico ed occupazionale di cui oggi abbiamo veramente bisogno.

la Lega Nord è da sempre vicina al mondo dell'agricoltura e fin da subito ha accolto con favore, tale provvedimento credendo nel mondo dell'agricoltura, da sempre parte sostanziale e predominante della nostra economia. Abbiamo accolto con favore questo provvedimento ed abbiamo cercato anche di dare il nostro contributo con alcuni emendamenti. Abbiamo appoggiato diverse proposte*, in primis* quella relativa al

e garantire che i prodotti arrivino a lieto fine. Abbiamo poi presentato un ulteriore emendamento per la semplificazione e la riduzione della burocrazia per quanto riguarda il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti; questo era un problema molto sentito da diversi anni, che attanagliava soprattutto le piccole e le medie aziende, che sappiamo tutti sono

Buona, anzi oserei definire ottima, l'iniziativa del Ministro: sta affrontando tutti i problemi in modo nuovo, oserei dire dinamico e propositivo ed i risultati si sono visti e si stanno vedendo, credo in maniera dirompente; penso che gli ultimi risultati che si sono ottenuti in quel di Bruxelles ne siano sicuramente una cartina di tornasole notevole. è sicuramente un problema che i precedenti Governi avevano cercato di risolvere. È un problema che si trascinava ormai da anni, ma che il nostro ministro Zaia e tutto il Governo hanno affrontato di petto e penso che i risultati ottenuti, come dicevo prima, si commentino

anche per il controllo forte e costante della qualità dei nostri prodotti; la loro promozione è sicuramente un valore aggiunto, ma anche la

all'estero. Se vogliamo affrontare di petto questa crisi, dobbiamo migliorare la nostra agricoltura su questo territorio, migliorando la credibilità dei nostri prodotti all'estero in modo che i nostri mercati possano espandersi in maniera forte e decisa. L'azione di questo Governo è un'azione che procede assieme agli agricoltori. I nostri agricoltori sanno che il ministro Zaia, tutto il Governo e tutti noi stiamo lavorando insieme a loro. Per questo motivo, la Lega Nord esprime un voto favorevole

onorevoli colleghi, non è il caso che io riprenda le questioni specifiche e i singoli temi che hanno costituito in questa sede oggetto di approfondimento e che hanno occupato, nella giornata di ieri e di oggi, la nostra attenzione durante la discussione generale sul decreto-legge in questione e durante la votazione degli emendamenti. Mi limiterò soltanto a ribadire un concetto concetto più volte evidenziato dai miei colleghi e dal sottoscritto, per conto del Gruppo del Partito Democratico, ma anche da diverse e qualificate espressioni della maggioranza, alla stregua delle analisi rese negli ultimi giorni da autorevoli fonti. Anche l'agricoltura italiana, che erroneamente si riteneva pressoché indenne, è interessata al fenomeno generale della recessione economica. necessiterebbero interventi, iniziative, sostegni concreti, affidamenti finanziari per tentare di risollevarne le sorti e rilanciarla. Quale migliore occasione della conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti per il rilancio - appunto - competitivo del settore agroalimentare? Noi senatori del Partito Democratico abbiamo colto appieno il senso di tale opportunità e ci siamo generosamente spesi nella predisposizione di alcuni importanti emendamenti, dialogando in spirito costruttivo con le rappresentanze dei Gruppi parlamentari di maggioranza in 9a Commissione e mettendo in campo un apporto assolutamente concreto, capace di intercettare le reali esigenze del comparto agricolo e le istanze più avvertite dalle categorie professionali e dalle forze sociali. un atteggiamento responsabile, volto a inviare un segnale corale ai settori in sofferenza: un segnale che costituisse un serio antidoto alla crisi che li attanaglia. In 9a Commissione si è stabilito un buon clima, come tanti di noi, a partire dal relatore senatore Piccioni e dal presidente Scarpa Bonazza Buora, abbiamo poi commentato intervenendo in quest'Aula. Eravamo, noi del Partito Democratico,

In rapida successione sono trapelate indiscrezioni, poi rivelatesi fondate, di bocciature da parte del Governo, e quindi della Commissione bilancio, anche di emendamenti favorevolmente e unanimemente licenziati dalla Commissione agricoltura: emendamenti, Qui si coglie il dato politico di una sostanziale chiusura della maggioranza ad ogni ipotesi di contributo delle opposizioni che comporti una ancorché minima revisione della linea del Governo, anche quando questa penalizzi settori vitali dell'economia italiana come l'agricoltura, il settore agroalimentare, la pesca (sulla quale avevamo centrato alcune azioni tese al riposizionamento e alla ristrutturazione delle imprese). Peraltro, eravamo incoraggiati a confidare in un ben diverso esito, dopo la dichiarazione del Presidente del Gruppo del Popolo della Libertà, senatore Maurizio Gasparri, riportata in una nota

al Senato il Gruppo PdL sta lavorando per risolvere una serie di questioni verso le quali il Governo ha mostrato la sua disponibilità. In particolare stiamo operando per recuperare risorse e proseguire nel rilancio del settore agricolo, oltre a trovare soluzioni a partire dalla fiscalizzazione degli oneri sociali e dagli interventi assicurativi. Si tratta di misure sulle quali ci auguriamo ci sia ampia convergenza e che, accanto alle iniziative già assunte dal Governo, quale la stabilizzazione dell'IRAP in agricoltura all'1,9 per cento, possano contribuire allo sviluppo di un settore fondamentale per la nostra economia». Malgrado un così autorevole pronunciamento della vigilia, il lavoro in Commissione, basato su un confronto leale dagli esiti praticamente unitari, è stato vanificato dal *diktat* del Governo e dalle conseguenti chiusure della maggioranza. Un'autentica falcidie delle proposte dell'opposizione, come ha appena rilevato anche il collega Di Nardo, di quelle della stessa maggioranza e di quelle congiunte, con un'unica eccezione, già modesta, poi ulteriormente immiserita dal fuori programma di un balletto di cifre. La compostezza con cui vi abbiamo assistito e persino il nostro voto favorevole al relativo emendamento, come gesto di attenzione - starei per dire di solidarietà - al mondo agricolo, non modificano il nostro giudizio su un risultato gramo. Parlo naturalmente del Fondo di solidarietà nazionale: il parere della 5a Commissione, che la Presidenza dell'Assemblea aveva annunciato come ostativo sull'intero emendamento, è stato poi corretto, ma in rapporto al solo primo comma; in merito alla dotazione richiesta di 200 milioni di euro per il triennio 2009-2011, ma soltanto per il 2008 e non per i 70 milioni di euro previsti dalla prima formulazione, ma per 65 milioni di euro. Abbiamo anche assistito - e concludo, signora Presidente - a qualche guizzo di teatralità da parte di qualche collega della maggioranza, nel tentativo, un po' scoperto, di depistare l'attenzione dell'Assemblea e di mascherare l'imbarazzo. Lo stesso ministro Zaia non si è sottratto - per così dire - quando ci ha intrattenuti sulle risultanze del negoziato sulla PAC, presentandoci l'argomento senza esserne richiesto, con la consueta enfasi che in quel caso non è giustificata. A seguito delle brusche virate, che solo in parte ho precedentemente accennato, con una maggioranza costretta a votare contro se stessa, si è formato un provvedimento disorganico, incapace di una seria risposta alla delicata fase congiunturale, del tutto insoddisfacente, che disillude le legittime aspettative dei settori interessati e che pertanto non può trovare partecipe il Gruppo del Partito Democratico, che per mio tramite preannuncia, infatti, il proprio voto contrario. Signora Presidente, onorevoli colleghi,

Questa è la prima considerazione che mi sento di fare. La seconda è di profondo rispetto e di infinito attaccamento - se mi è consentito - alla Commissione che ho l'onore e il privilegio di presiedere.

alla difesa e alla propugnazione più attiva e utile possibile del settore che ci è stato affidato. È, quindi, assolutamente vero quello che diceva ora il collega, ministro ombra, senatore Andria, a nome del suo Gruppo;

che si tratta di un provvedimento che è stato caricato di troppe attese. Mi sento, quindi, di confermare in pieno la dichiarazione che veniva citata poc'anzi dal collega Andria e attribuita assolutamente correttamente, penso, al Presidente del Gruppo cui appartengo,

anche in questa occasione perché il provvedimento potesse avere la maggior sostanza possibile compatibilmente con i vincoli di bilancio. Voglio ricordare a me stesso, senza andare a ripercorrere in maniera pedissequa tutto quanto è stato fatto e ottenuto,

e all'importante lavoro svolto dal relatore Piccioni, risultati significativi come, per esempio, la conferma del fondo di solidarietà nazionale, cioè delle assicurazioni agevolate per gli agricoltori per il 2008

che permetteranno al Governo di poter trasferire agli agricoltori risorse significative per coprire il finanziamento agevolato delle assicurazioni per l'anno 2009. Gli agricoltori italiani, quindi, non devono essere tratti in inganno, nessuno l'ha voluto fare, me ne rendo ben conto: i soldi per le assicurazioni ci sono per il 2008 e per il 2009. Questo è un risultato, secondo me, significativo. Per quanto riguarda le agevolazioni previdenziali, con grandissimo sforzo da parte del presidente Azzollini e della sua Commissione é stato raggiunto un significativo risultato che porta al 31 marzo prossimo la proroga delle agevolazioni. Naturalmente serviranno dal Sottosegretario, che né è assolutamente consapevole - un nuovo decreto e un nuovo provvedimento prima del 31 marzo prossimo perché evidentemente questa è un'iniziativa legislativa che deve assolutamente durare. Per quanto riguarda l'ICI sui fabbricati rurali, voglio sommessamente ricordare ai colleghi del centrosinistra che la nuova disciplina dell'ICI sui fabbricati rurali è stata introdotta - dico questo non per fare un rimbalzo di responsabilità - dal vostro Governo precedente; é stata una misura del vice ministro dell'epoca Visco, che è stata poi applicata in un modo un po' stravagante da parte dell'amministrazione competente. Dunque, io credo che ci sarà lo spazio - il ministro Zaia ieri ce ne ha dato conferma e il Sottosegretario è qui a testimoniarlo

Sono state fatte importanti semplificazioni nel settore dell'agricoltura e della pesca. Per quanto riguarda la pesca, senatore Andria, ricordo a me stesso che è in elaborazione presso la nostra Commissione un disegno di legge che porta la mia firma e sul quale tutti quanti noi potremo esercitarci, penso e spero con profitto, per portare a casa quei risultati attesi dal mondo armatoriale da un lato e dal mondo della cooperazione, della pesca e dell'acquacoltura italiana. Quindi, in sostanza, colleghi, io credo che,

sono inseriti i seguenti: ". Si tratta soltanto di un'operazione di *drafting*, Presidente.

poiché la 7a Commissione non ha concluso l'esame del disegno di legge sull'università, la discussione avrà luogo nella seduta antimeridiana di domani. Ricordo che domani pomeriggio, alle ore 15, si svolgeranno, con trasmissione in diretta televisiva, interrogazioni a risposta immediata immediata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulle infrastrutture nel Mezzogiorno, con particolare riguardo al ponte sullo stretto di Messina. Durante lo svolgimento del sindacato ispettivo in Assemblea, le Commissioni sono autorizzate a proseguire i propri lavori. A conclusione delle interrogazioni a risposta immediata, la seduta dell'Aula sarà sospesa e riprenderà, come previsto dal calendario dei lavori, alle ore 17, con il seguito degli argomenti all'ordine del giorno.

desidererei richiamare l'attenzione dell'Aula sui tragici fatti e sulle vittime delle inondazioni che hanno colpito il Brasile, fatto di grande gravità che richiede l'attenzione di quest'Aula. Le inondazioni che stanno colpendo lo Stato di Santa Caterina, dove c'è una forte e radicata presenza di immigrati veneti, non possono lasciarci indifferenti come sembra invece che accada Colleghi, stiamo parlando di persone morte e di milioni di sfollati. Gli sfollati sono circa un milione e mezzo, il numero dei morti è salito a 100, è ancora in crescita e il bilancio potrebbe aggravarsi dato che alcune città sono ancora isolate e le condizioni meteorologiche peggioreranno nel corso delle ore e nei prossimi giorni. Le città maggiormente colpito sono Itapoà, Benedito Novo, Rio dos Cedros, Pomerode e Blumenau, località in cui è molto forte la presenza dei nostri emigrati di terza e quarta generazione.